del processo verbale della seduta pomeridiana del 24 marzo*.

il provvedimento che ci accingiamo ad affrontare, il disegno di legge n. 2568, già presentato l'8 marzo scorso in quest'Aula e successivamente rinviato in Commissione giustizia, torna nuovamente all'esame dell'Assemblea. Dopo ulteriori approfondimenti in Commissione, dove si sono tenute anche una serie di audizioni che hanno consentito di comprenderne meglio i molteplici aspetti, abbiamo ritenuto abbiamo ritenuto opportuno lasciare il testo del disegno di legge intatto, così come è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, e di proporne l'approvazione definitiva in questa sede, senza apportare quindi ulteriori modifiche. anche alla luce del fatto che, dopo questo ulteriore attento esame, i ritocchi e le correzioni pensati e in grado di essere approvati si sono rivelati marginali, quindi in numero esiguo e non così essenziali da costringere ad un ritorno all'esame della Camera. Su alcune proposte emendative, oggetto di discussione in sede di Commissione, sono state espresse diverse perplessità. Molti emendamenti minano la funzione discrezionale del giudice; altri non presentano i requisiti della copertura finanziaria (a tal proposito ricordo anche il parere contrario della 5a Commissione); tutti gli altri non giustificano il rinvio del provvedimento alla Camera. In buona sostanza, tale decisione è da ricondurre all'importanza - proprio all'importanza - che tutti noi attribuiamo a questo provvedimento e quindi alla necessità di una sua celere approvazione, evitando un suo procrastinarsi che rischierebbe di essere a tempo indeterminato. Ci saranno sicuramente momenti successivi all'interno dei quali rafforzare l'intervento. II provvedimento è essenziale in quanto non solo affronta nuovamente, con la finalità di potenziarli, i diritti che vanno riconosciuti alle donne madri in stato di detenzione ma, soprattutto, cerca di consolidare le tutele inalienabili dovute avanti a tutto, prioritariamente, ai figli minori di queste donne. L'obiettivo di questo provvedimento - lo ricordo, cari colleghi - è quello della tutela del minore ed è anche la prima risposta concreta a una volontà espressa non molto tempo fa dal ministro guardasigilli Alfano, che disse: «Mai più bambini in carcere». Si tratta certamente di una volontà condivisa da tutti. Parliamo di una legge di buonsenso che rientra nella più ampia cornice dei diritti delle donne, ma soprattutto dei minori e che assicura ai bambini di crescere, nonostante la loro particolare e non felice condizione, in strutture adeguate, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza a cui sono sottoposte sottoposte le loro madri: perchè una proposta di taglio così civile non deve però indurre, cari colleghi, ad una interpretazione non corretta, in quanto riteniamo fondamentale, allo stesso tempo, il principio della certezza della pena. Il provvedimento è stato concertato in modo tale da consentire garanzie a tutela per i reati gravi. Non cerchiamo affatto di ridurre surrettiziamente l'impatto deterrente delle sanzioni per le donne che commettono reati solo perché madri. Per quanto concerne invece la questione della visita da parte delle madri detenute ai minori ricoverati che tanto ha acceso la discussione, di fatto è protetta dall'esistenza di una clausola di salvaguardia da parte dell'ordinamento e all'interno dello stesso provvedimento. E comunque, confidiamo nel giudice e nella giurisprudenza. Non si tratta di un provvedimento bandiera, né tantomeno di un provvedimento manifesto: è piuttosto una tappa fondamentale per proseguire nell'azione di tutela dei minori. Certo, ora più che mai, e mi rivolgo all'Aula tutta, ai colleghi di maggioranza e di opposizione, è importante accelerare la realizzazione delle forme attenuate di detenzione, come quella che già esiste a Milano, che sicuramente avranno un impulso fortissimo dall'approvazione immediata di questo provvedimento.

Signor Presidente, stamane mi sono recato a Milano a visitare l'unico istituto di custodia attenuata per detenute madri esistente in Italia (tra l'altro, uno dei pochi in Europa), che dipende dal carcere di San Vittore. Ho potuto ammirare, perché in effetti si ammira, l'applicazione della nostra Costituzione. È un istituto, creato nel 2006 ed entrato in funzione nel 2007, con 16 madri e altrettanti bambini.

Cosa c'è nella legge che oggi ci apprestiamo ad affrontare che potrebbe migliorare questa situazione? Forse, e dico forse, soltanto un particolare: si eleverebbe l'età dei bambini che possono stare con il loro genitore - ahinoi nella legge si insiste ancora soltanto nella possibilità per la madre di poter restare con i propri bambini - dai tre ai sei anni,

annunciare una serie di misure, salvo poi non mantenere neanche la promessa dell'annuncio e, quando si va a vedere che cosa è stato annunciato, scoprire che nei dettagli si insinua il diavolo.

quando si vanno a interpellare, ancora una volta, i rappresentanti del Ministero della giustizia, non si riesce ad avere una lista certa e definitiva di quali siano le Istituzioni che in effetti partecipano. Si vocifera di ICAM a Venezia, a Firenze e a Roma, ma, parlando anche con la controparte (molto spesso la Regione, che dovrebbe dare in comodato d'uso alcuni locali) non si riesce a capire se in effetti tutto ciò sia stato firmato e, se firmato, quali siano i tempi certi della consegna della struttura stessa.

questi processi di ratifica di convenzioni perché entro il 2011 (se possibile, quindi, a un anno dall'adozione di questa misura) si possano finalmente avere degli istituti a custodia attenuata per le detenute madri (e, si spera, anche per i detenuti padri) e anche

questo provvedimento, uscito - ahinoi - con la quasi unanimità dalla Camera, perché la delegazione radicale non ha partecipato al consenso che si è creato attorno ad esso, come fosse un qualcosa che va a migliorare la condizione delle detenute madri. Abbiamo presentato molti emendamenti, ma credo che lo scetticismo circa la novità o l'ulteriore aiuto ai bambini (e non - ricordiamolo - alle detenute madri) contenuto in questo provvedimento, vi sia realmente. Su questo torneremo più avanti, anche con la senatrice Poretti, con una serie di emendamenti, che credo Concludo con una nota di metodo. Siamo arrivati molto velocemente al dibattito in Aula tre settimane fa ed è stato concesso un ritorno in Commissione di due settimane, per poi arrivare, alla fine di audizioni molto importanti e formative (oltre che informative), alla decisione che le modifiche potevano essere solo due: concedere la possibilità di visitare più a lungo i figli in ospedale e modificare il titolo del provvedimento. Se questa è la disponibilità del Governo, non ci si venga poi a lamentare che esistono delle insistenze su alcune questioni fondamentali di principio, *in primis* il rispetto della nostra Costituzione.

Restava in sospeso la presenza del ministro Maroni in quest'Aula per riferire sulla vicenda che riguarda Lampedusa. Apprendiamo da agenzie che il ministro Maroni avrebbe

non solo al ministro Maroni, ma anche al ministro Galan - la disponibilità a venire in Aula al Senato. Nel momento in cui, nel corso di questa seduta, sarà fatta una comunicazione ufficiale

tra detenute madri e figli minori, e lo facciamo a distanza di non molti giorni da quando abbiamo affrontato in quest'Aula la discussione generale ed abbiamo poi deciso di rinviare il testo del disegno Come ci ha ricordato anche la relatrice, siamo oggi a votare lo stesso testo che è stato approvato quasi all'unanimità dalla Camera

grazie. secondo il nostro ordinamento e secondo un principio di giustizia sacrosanto, devono scontare la pena in carcere, con la conseguenza che i loro figli sono costretti a vivere i primi anni di vita dietro le sbarre. Secondo il Secondo il sistema attualmente vigente nel nostro ordinamento, madri e figli vivono all'interno degli istituti di pena in appositi spazi denominati «asili nido»,

Gli spazi all'interno del carcere chiamati «asilo nido» conservano invece tutte le caratteristiche del carcere, e quindi sono sottoposti allo stesso regime di vigilanza e di sorveglianza.

Sono privati anch'essi della libertà, oltre che di quegli slanci, di quegli atteggiamenti e movimenti che sono tipici della loro età e dei loro coetanei, che hanno invece la fortuna di vivere all'interno di nuclei familiari. Le statistiche accreditate dimostrano che questi bambini soffrono, per esempio, di inappetenza e di apatia, oltre che di gravi disturbi legati al sovraffollamento e alla mancanza di spazio; sviluppano inoltre dei problemi di comunicazione e di relazione, che pregiudicheranno purtroppo in modo significativo la loro crescita. Una simile situazione non può essere arginata sottraendo i minori alle loro madri, perché in questo modo i bambini verrebbero privati dell'affetto più importante, che è quello di una madre: di una madre che ha sbagliato agli occhi della società, e che quindi è giusto che sconti la sua pena, grazie.

Alcuni studi dimostrano infatti che un figlio allontanato dalla madre, perché costretta a scontare una pena in carcere, è un soggetto vulnerabile, potenzialmente più esposto rispetto ad altri coetanei ad avere in futuro problemi con la giustizia e quindi a reiterare l'errore. Per migliorare questo triste scenario diventa dunque fondamentale prevedere tre misure, che sono quelle contenute in questo disegno di legge: introdurre ipotesi alternative alla detenzione negli istituti di pena; migliorare le condizioni della detenzione nelle carceri; estendere l'applicabilità dell'istituto degli arresti domiciliari in favore delle madri con figli minori. Il provvedimento si dirige proprio in questa direzione e possiede un importantissimo valore storico e normativo. La lente attraverso la quale dobbiamo leggere le disposizioni in esame è quella della garanzia del diritto di ogni bambino ad una crescita sana, giusta ed equilibrata. Dico questo per evitare la nascita di opinioni e interpretazioni che tradirebbero la *ratio* ispiratrice di queste norme. L'introduzione e la diffusione dei cosiddetti Istituti a custodia attenuata e la possibilità di scontare gli arresti domiciliari in una casa famiglia non dovrebbero essere intese come un beneficio attribuito *tout court* alle detenute in contrasto con il principio della effettività e della certezza della pena: tutt'altro. Con queste disposizioni non si sottraggono le donne alla pena del carcere, azzerando la sentenza di un giudice, né si introduce a livello generale una causa di esclusione dalla pena legata alla condizione di madre di una detenuta. Guardando invece il tutto dalla giusta prospettiva, emerge che questo provvedimento offre la possibilità di scontare la detenzione in strutture consone ad un minore e alla dignità umana, per evitare che siano i figli le uniche vittime del sistema punitivo. È doveroso ricordare che l'articolo 27 della nostra Costituzione stabilisce che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Io non vedo quale rieducazione o riabilitazione possa scaturire da una situazione in cui una donna veda giorno dopo giorno, nello sguardo del figlio innocente, gli effetti del suo debito con la giustizia. Non reputo neppure che la convivenza dietro le sbarre di un carcere costituisca un trattamento conforme al senso di umanità, secondo quanto prescritto dalla nostra Carta fondamentale. Un moderno Stato democratico e di diritto dovrebbe essere dunque in grado di coniugare la certezza della pena con l'umanità e dignità per figli delle detenute. Entrando nel merito delle disposizioni normative, valutiamo positivamente l'innalzamento da tre a sei anni dell'età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere. Qualora non sia possibile evitare la custodia cautelare, si introduce la possibilità di scontare questa misura non più in carcere, ma in un Istituto a custodia attenuata per detenute madri, conosciuto con il nome di ICAM. ICAM. Un'ottima struttura ormai consolidata negli anni, che può essere mutuata su tutto il territorio nazionale e che produce effetti positivi sia sul bambino sia sulla madre detenuta che deve scontare la pena è stata realizzata a Milano. È una struttura che non ricorda in alcuna maniera il carcere, essendo simile a un asilo nido vero, dove per esempio gli operatori della polizia penitenziaria lavorano senza divisa; di spazi ben areati e luminosi, dove il bambino immagina e vive l'esperienza di una casa dove poter stare con la propria madre. Altra rilevante novità è l'introduzione di una norma di carattere generale che introduce invece la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso una casa famiglia protetta. Si tratta di una concreta alternativa per le donne, soprattutto straniere, che hanno commesso dei reati, che però non possiedono un'abitazione in cui scontare gli arresti domiciliari. Quindi offriamo una soluzione anche a questa tipologia di detenute. Degne di nota sono anche le disposizioni che introducono il diritto di visita al minore infermo e il diritto di assistere il figlio durante visite specialistiche resesi necessarie in relazione a gravi condizioni di salute.

un tempo, quindi, eccessivamente lungo, sarebbe, invece, stato opportuno anticipare tale termine per consentire una più immediata applicazione delle misure ivi previste.

e la libera volontà di vivere la vita nel modo in cui desideri farlo. Tutto il resto lo prendiamo soltanto in prestito». Noi oggi, approvando questo provvedimento, possiamo restituire ai figli delle donne detenute in carcere la dignità sociale che credevano perduta e soprattutto la possibilità per loro di continuare a sognare. Quindi, pur con alcune parti non del tutto corrette, credo che questo provvedimento debba essere al più presto approvato.

di illustrarlo) scaturisce da una nostra recente visita - mia e di alcuni colleghi dell'Italia dei Valori - alla casa circondariale femminile di Rebibbia di Roma. Rebibbia, come sapete, rappresenta già un buon carcere, che possiamo annoverare tra le strutture modello del nostro Paese,

sia sotto il profilo del numero di detenute in relazione alla capienza, sia sotto quello della dotazione del personale. Tralascio i dati relativi al sovraffollamento della struttura e quelli relativi alla carenza di organico passo subito alle nostre richieste, che speriamo vengano benevolmente accolte da quest'Assemblea. Chiediamo al Governo di assumere le opportune iniziative volte a colmare con urgenza le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie in generale e delle case circondariali femminili in particolare, reperendo i fondi necessari per completare l'organico degli operatori penitenziari, compresi psicologi ed educatori, e provvedendo anche alla stabilizzazione delle lavoratrici precarie e delle puericultrici in particolare, in considerazione anche della loro peculiare esperienza. Chiediamo di disporre opportune verifiche all'interno degli istituti al fine di accertare se le condizioni strutturali e le risorse economiche e umane disponibili siano tali da assicurare l'attuazione del diritto al lavoro in carcere, sulla base delle positive esperienze già registrate in tanti Paesi europei. Chiediamo infine di reperire idonee risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retributivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, nonché per l'edilizia penitenziaria, prevedendo la realizzazione di nuove strutture ove necessario e dando priorità all'ampliamento e all'ammodernamento di quelle esistenti. Tutto ciò chiediamo con urgenza, per migliorare davvero le condizioni di vita nei penitenziari, e dei detenuti e degli operatori, che vi lavorano davvero con grande professionalità, perché davvero possiamo rispondere al richiamo dell'articolo 27 della Costituzione alla funzione rieducativa della pena. *(Applausi

Di nuovo c'è poco da dire. Siamo convinti che serva una legge di grande umanità quale questa: una legge che, dal momento che c'è un bambino in gioco, ne tuteli l'esigenza di vivere con la madre, al punto da attenuare e sospendere eventuali misure cautelari o condanne subite dalla stessa.

i figli non dovrebbero pagare per colpe non loro, dovrebbero poter crescere nel migliore ambiente possibile. Quello che prevede la norma, infatti, è che anziché in carcere le pene possano essere scontate in ambienti più idonei e adatti alla crescita dei figli: case protette, istituti a custodia attenuata, fino ad arrivare agli

Quando scriviamo che possono assistere i figli non solo le madri ma anche i padri qualora queste si trovino in gravi condizioni di salute, non possiamo non pensare che, trovandoci in questo Paese, dove abbiamo visto un po' di tutto, un certificato o un referto medico un tantino adeguati allo scopo dovremmo anche metterli in preventivo. Stante che in carcere si va anche troppo poco, se si offrissero troppi spazi alternativi o vie di fuga rischieremmo di compromettere effettivamente il senso della giustizia. Infatti, come Lega, ci troviamo un tantino imbarazzati tra l'approvare una norma che introduce una certa umanità nello scontare la pena e il rischio di vanificare il senso della giustizia oppure anche la certezza della pena.

degli assistenti sociali che esprimono giudizi di non idoneità o di non adeguatezza, o trovano qualche disturbo nelle madri, al punto da allontanarle dal proprio figlio. Questi sono veri e propri drammi, perché si rovinano la vita non solo dei figli

Una madre, magari sola, che perde il posto di lavoro si trova probabilmente in grandissime difficoltà anche a pagare l'affitto della casa; non pagando l'affitto della casa, normalmente subisce un provvedimento di sfratto costretta a trovare situazioni alloggiative di fortuna e se, in quel momento, arriva una valutazione non appropriata di un assistente sociale può vedere addirittura revocare la potestà genitoriale. Il tutto parte da situazioni di carattere economico. Ben venga questa normativa che attutisce le pene,

Ci dispiace che il lavoro svolto in Commissione non abbia prodotto le modifiche che sarebbero state necessarie.

superiore delle persone minori di età, in particolare al di sotto dei tre anni, vivono momenti di fragilità. Se poniamo al centro del nostro ragionamento

base imprescindibile per poter crescere e sviluppare le proprie potenzialità. Ma tale diritto alla relazione va assicurato in modo ancora più forte laddove le persone minori d'età, in particolare al di sotto di tre anni, siano colpite da malattia.

per reati non commessi. Noi dobbiamo sapere, quindi, che «il più possibile» significa: mai custodia cautelare per le madri detenute, custodia attenuata e, soprattutto, case famiglia. In questo caso, il provvedimento in esame ci colpisce perché non ha risolto alcune delle grandi questioni sollevate dal dibattito

L'articolo 4 demanda a un successivo decreto ministeriale i requisiti che le cosiddette case famiglie protette debbono possedere, lasciando incertezza sulle loro modalità di gestione e di realizzazione. Così facendo, si corre il rischio che anche in queste famiglie l'elemento di sicurezza finisca per prevalere sulle esigenze educative del minore. Per questo motivo in tutto il testo normativo abbiamo proposto la soppressione della parola «protette», associata alle case famiglie, proprio a dimostrazione del fatto che in queste strutture l'elemento di tutela della sicurezza deve necessariamente essere contemperato con le esigenze educative del minore. Per quanto attiene alla copertura, sia per gli istituti a custodia attenuata che per le case famiglie, infine, attenuata che per le case famiglie, infine, si prevede una copertura finanziaria assolutamente insufficiente. Quanto alle seconde, l'articolo 4 prevede la possibilità di realizzare queste strutture previa convenzione con gli enti locali, senza però oneri aggiuntivi. Per quanto riguarda invece gli istituti a custodia attenuata, vi è nell'articolo 5 una clausola di compatibilità con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto, che rischia di rendere minime le risorse a disposizione.

Nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la custodia cautelare deve essere eseguita in un istituto a custodia attenuata. In mancanza di posti sufficienti presso gli istituti a custodia attenuata, il nuovo comma 2 dell'articolo 285*-bis* stabilisce che la misura debba essere eseguita presso case famiglia. Abbiamo, infine, anticipato il momento di entrata in vigore della norma al gennaio 2012. Quanto all'articolo 2, sono state proposte da noi delle modifiche, volte a garantire che la madre possa assistere con continuità il minore ricoverato in gravi condizioni di salute. Il termine «visitare» riferito all'infermo è stato sostituito con la parola «assistere», proprio per esplicitare che la madre deve poter stare in ospedale con il proprio bambino per tutta la durata del ricovero, e non solo in occasione di sporadiche visite. Ad ulteriore garanzia di una interpretazione non equivoca della norma, si è indicato in maniera espressa che la durata dell'assistenza della madre non può essere inferiore al periodo di ricovero del bambino e, comunque, non può cessare fino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi. È stato infine aggiunto un comma 3 che consente alle madri, che siano detenute assieme ai loro bambini minori di tre anni, di assistere i figli negli eventuali ricoveri presso strutture extrapenitenziarie, a prescindere dalla gravità delle condizioni di salute. Per il bambino che vive assieme alla madre, infatti, la mancanza del genitore convivente in un momento di difficoltà avrebbe comunque effetti traumatici, a prescindere dalla gravità della patologia. L'articolo 3, infine, è stato da noi modificato al fine di escludere in ogni caso che le condannate, madri di bambini di età inferiore a 10 anni, scontino la loro pena in istituti ordinari. Per quanto riguarda il comma 1-*bis*, è stato eliminato il riferimento all'articolo 4-*bis* e si è stabilito che la quota di pena necessaria per accedere al beneficio in esame debba (e non possa)

che riguardano il tema della giustizia e della pena. Con l'ordine del giorno G202

si occupi della riorganizzazione del momento punitivo limitando il ricorso alla pena detentiva. Come è noto e come peraltro è stato più volte

un minore onere a carico dello Stato e con una maggiore capacità di recupero di chi sconta questo tipo di pena.

anche un risparmio enorme rispetto al costo che la traduzione di un detenuto comporta.

riguarda l'opportunità di adottare iniziative volte ad individuare ed elencare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza cui fa riferimento il provvedimento. Rispetto a questo ordine del giorno ho avuto un'interlocuzione con la sottosegretario

signor Presidente, l'ordine del giorno G205, che mira ad estendere le previsioni riguardanti la realizzazione di strutture destinate alle detenute madri anche ai detenuti padri che si trovano nelle medesime condizioni. L'intero provvedimento peraltro è così concepito, ma relativamente alla

Il testo origina - come è noto e come è stato sottolineato da tutti quelli che anche oggi sono intervenuti in Aula - dalla necessità di apprestare un'adeguata tutela ai diritti universalmente tutelati tutelati dei genitori e dei figli, rispetto ai quali le differenti posizioni politiche non possono che convergere. I problemi che nascono nel rappresentare la situazione della donna detenuta sono dovuti al fatto che la realtà delle carceri è stata creata e pensata nelle strutture, nelle regole, nelle relazioni, nel vissuto da e per gli uomini. L'universo detentivo femminile viene visto attraverso una prospettiva unicamente maschile che ha, quindi, profonde difficoltà a cogliere gli aspetti di specificità e tipicità propri delle donne, che la detenzione, al contrario di quanto si possa comunemente credere, non cancella, ma anzi rafforza. E, senza alcun dubbio, la questione principale che la detenuta porta con sé è quella determinata dalla maternità e dal difficile rapporto che viene ad instaurarsi tra le madri-detenute e i propri bambini, i quali vengono sottoposti al trauma psicofisico di vivere dietro le sbarre con le proprie mamme subendo, quindi, forti e profondi limiti nello sviluppo della propria personalità. Prevedere una pena che divida traumaticamente una donna dal figlio o permetta loro di essere uniti solo in condizioni di restrizione rappresenta senza alcun dubbio una soluzione disumana, grava non soltanto sulla detenuta madre, ma anche sul figlio. Con l'odierno disegno di legge si intende affermare con forza il rispetto di un principio di alta giustizia e di grande umanità, attuando concretamente uno dei doveri della Repubblica, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che consiste nel rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità, nel caso di specie la personalità del figlio la cui madre sia sottoposta a misure cautelari o a un provvedimento restrittivo della libertà personale. La *ratio* dell'odierna proposta legislativa è particolarmente apprezzabile, posto che, oltre a tutelare in via preminente l'interesse del minore ad un corretto sviluppo psicofisico, si inserisce nell'ambito dei provvedimenti che prevedono l'attribuzione di un'adeguata rilevanza giuridica alle misure alternative alla detenzione, riuscendo a coniugare due diverse esigenze: quella della tutela del rapporto tra la madre detenuta e il figlio minore e quella della sicurezza. Proprio le osservazioni critiche emerse nel corso della discussione in Aula rappresentano, a mio avviso, un punto di forza del provvedimento. Lasciare la decisione alla discrezionalità del giudice, anziché tipizzare le ipotesi di reato, non significa necessariamente restringere il campo dei benefici concessi alle detenute madri. È al contrario una garanzia per le mamme e per i loro bambini, dal momento che chi giudica gli strumenti e la sensibilità per valutare i singoli casi. A ispirare questa scelta, quindi, è la convinzione che il giudice saprà orientare la sua decisione seguendo un unico punto di riferimento: la condizione migliore per i bambini. Pure sul fronte - anche oggi sollecitato - dei ricoveri ospedalieri dei minori, richiamarsi al concetto di assistenza è vago. Preferiamo sia il giudice a fissare tempi e modalità dei permessi, senza precludere alle madri la vicinanza ai loro figli ammalati, da un lato, e senza tralasciare le esigenze di vigilanza del sistema penitenziario, dall'altro. La possibilità di ricreare all'interno delle strutture penitenziarie un ambiente più adatto ai bambini, senza divise, tintinnio di chiavi, sbarre e porte blindate, sulla scia dell'esperienza dell'ICAM di Milano, rappresenta, infatti, il cuore del provvedimento, insieme all'opportunità di ospitare le detenute madri e i loro piccoli in case famiglia. La permanenza più lunga (fino a sei anni) dei figli con le mamme è un altro passo nella direzione di una corretta crescita del minore che, inoltre, in caso di pericolo di vita o, comunque, in gravi condizioni di salute, potrà contare sulla presenza della madre in ospedale: alla detenuta o imputata si concede il permesso di recarsi nei nosocomi per assistere il proprio bambino. Con il testo oggi sottoposto al vostro voto si intende dare un ancor più completo riconoscimento alle conquiste culturali ottenute dalle donne negli ultimi quarant'anni, a cui, insieme con i principi di legalità e uguaglianza, si intende e uguaglianza, si intende collegare una forte enfatizzazione dei legami parentali - tra i quali fondamentale valore ricopre, naturalmente e doverosamente, quello esistente tra madre e figlio - che per ottenere una compiuta realizzazione devono essere sostenuti, come avviene nel caso di specie, da condizioni Per tutto questo, auspico l'approvazione del disegno di legge. costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». Commissione affari costituzionali, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando, quanto agli emendamenti 3.200 e 3.202, che le disposizioni ivi previste, in materia dì predisposizione di case di accoglienza, presuppongono un necessario accordo con gli enti locali interessati». enti locali interessati». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.216, 1.218, 4.206, 4.0.200, 4.0.202 e 4.0.203. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.220, 1.223, 1.224, 1.225, 1.226, 2.202, 2.203 e 4.202. Esprime parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

entro il 2014 questa legge ha significato, altrimenti è solo una bandiera.

rivolgiamo il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di studio.

**Il Senato non approva.**

Dal momento che abbiamo tanto parlato di bambini che necessitano nelle carceri di assistenza, soprattutto sotto il profilo psicologico, ricordo che ci sono 39 psicologi

poi ci si è accorti che di femminile aveva ben poco, perché l'interesse protetto doveva prioritariamente essere quello del minore, e non tanto quello della mamma.

La legge del 1975, in epoca non esattamente reazionaria, aveva cercato di mediare tra queste esigenze e di trovare un punto d'incontro; noi, viceversa, stiamo superando tutto questo, introducendo delle ingessature ai criteri di pronunciamento dei magistrati, in particolare dei giudici di sorveglianza,

facendo solo questa considerazione di carattere sociologico, dovremmo semplicemente sopprimere la pena, non prevederla in alcun caso, senza ricercare dunque il punto di equilibrio tra queste differenti esigenze.

annullando il carattere restrizionale della pena e l'effettività della stessa. Ma questo non è un punto di vista reazionario: è una considerazione che all'atto pratico è evidente. Concludo su questo punto, facendo presente alla luce di quanto abbiamo lungamente discusso in Commissione, dove non ci siamo girati i pollici in queste due tornate dalla nostra Commissione giustizia. I casi di donne che si trovano in stato di detenzione sono tre.

la permanenza in carcere è soltanto di sei, otto mesi circa, come abbiamo sentito dalle statistiche. Ma il richiamo alla recidiva non esiste più? termini, mentre il magistrato di sorveglianza anche oggi ha la facoltà di valutare la pericolosità sociale in concreto, e se si tratta di reati minori che non suscitano allarme sociale può dare il beneficio, volete dire che comunque, astrattamente, sia opportuno privilegiare questo tipo di rapporto anche rispetto ad un caso - e non è scolastico - che veda, ad esempio, la genitrice commettere due reati, uno la mattina ed uno il pomeriggio, tutti della stessa indole (generalmente reati contro il patrimonio per la verità), e che questo escluda

quando la permanenza del rapporto madre-figlio è importante non solo per il figlio ma financo per la madre nella lettura rieducativa della pena detentiva. Ma qui non c'è alcuna distinzione di questo genere. Ecco perché la trovo una norma-manifesto, demagogica, che rischia di essere addirittura peggiorativa rispetto al funzionamento della vigente legge n. 354 del 1975, ed è questa la ragione molto semplice,

è tecnicamente ed organizzativamente un piccolo passo in avanti, e questa sarebbe l'unica cosa da salvare, obiettivamente a beneficio del sistema e delle persone e delle famiglie interessate, nell'articolo 1. *(Applausi dei

dei sei anni se la pena residua che la madre deve scontare è inferiore a sei mesi. Questo perché

che è stato dato parere contrario ai miei emendamenti, che sono stati pronunciati inviti al ritiro agli emendamenti presentati dai colleghi della Lega, che sono nei loro contenuti sostanzialmente equipollenti ai miei.

dall'onorevole relatrice e dall'onorevole Sottosegretario alcun invito al ritiro, mi contenterò di vedere respinti con sdegno i miei emendamenti, e li mantengo.

Camera; evidentemente il Senato non ha possibilità di intervenire, anche laddove verifica che vi sono degli errori e degli aspetti che sarebbe utile correggere.

cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

detenuti nelle carceri. Altrimenti, dobbiamo davvero interrogarci sull'utilità di questo consesso e di questa istituzione.

soddisfare le esigenze cautelari, e quindi le esigenze di tutela della collettività, e che allo stesso tempo consentono, a chi ne deve beneficiare, di avere una vita diversa da quella carceraria. Nel nostro ordinamento non è stata data mai attuazione alla norma sul braccialetto elettronico. Non comprendiamo per quale ragione questo non avvenga,

a non approvare se restano sotto i giornali, o le giacche, o pezzettini di carta,

Invito il senatore Di Nardo e la senatrice Vicari ad effettuare un controllo

Allora, rischio di trovarmi nuovamente solo in compagnia del buon senso. Quindi, siamo in due e rimaniamo isolatissimi: io ed il buon senso siamo isolati.

non ho timore della solitudine, quando sto con il buon senso. sta per approvare, respingendo anche il mio emendamento, una dicitura che vi leggo testualmente: «se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano». Voglio portarvi l'affettuoso ringraziamento da parte dei detenuti padri perché sono destinati a poter alloggiare in una casa a custodia attenuata destinata alle detenute madri che certamente

Basti pensare che il lessico che conoscono è quello carcerario e le prime parole che dicono sono quelle che sentono dire ai secondini. Le loro vite sono scandite come quelle dei detenuti, la loro vita all'aria aperta è confinata alle pochissime ore in cui qualche associazione di volontariato, se c'è, li porta fuori.

sarebbe se ci fosse il padre - per una loro crescita equilibrata. Stiamo parlando, cioè, di sofferenza, di privazione, di dolore, di mortificazione, di bambini. La spiritosaggine su questo aspetto, magari fondata su un testo mal scritto, francamente la trovo del tutto

Mi pare che su questo disegno di legge nessuno stia scherzando, tant'è che i disagi che sono stati adesso manifestati

colleghi del suo stesso Gruppo si sono dati cura, con il successivo emendamento 1.215, di fronteggiare

«La stessa disposizione si applica, presso uno specifico istituto a custodia attenuata» - il fatto che poi questo sia praticamente inattuabile è altro discorso, però i colleghi del suo Gruppo si sono posti il problema che ho segnalato - «, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia il padre». Come vede, ho evidenziato, sia pure in forma paradossale, ma che non è un caso di scuola, una situazione che colleghi del suo Gruppo, con i quali evidentemente lei non mantiene un rapporto minuto per minuto, come del resto è concepibile per il Presidente di un Gruppo così esteso,

verso la popolazione detenuta, verso l'opinione pubblica e verso la dignità intellettuale di noi legislatori, che nessuno di noi minimamente si è sognato di fare ironia su situazioni che non siano di per se stesse paradossali, e se, con ironia, alle volte si cerca di richiamare l'attenzione di un'Aula che altrimenti con discorsi seri risulta soltanto annoiata, e ti tacita e basta, questa è colpa collettiva di tutti noi, a cominciare da me, ma non certamente solo mia. Ad ogni buon conto, voglio sottolineare che in Commissione abbiamo lavorato per lunghe settimane su questo testo e che nessuno ha sottovalutato la gravità dei problemi che si pongono, del rapporto tra genitori e figli. Abbiamo anche detto che si tratta di arrivare ad un equilibrio tra questa esigenza e la tutela delle aspettative di chi ha madri, padri e figli che hanno subito la commissione di reati, anche gravi, e le conseguenze degli stessi. Ci sono infatti fior di nostri concittadini che hanno figli piccoli Grazie,

dopo averlo rinviato in Commissione è figlia di questo esame approfondito, e non di superficialità! PRESIDENTE.

Noi avevamo pensato di approfondire alcune tematiche per migliorare la legge e, soprattutto, per rendere più umano il trattamento delle detenute madri in funzione dei figli. L'interesse prevalente, quindi, era quello dei minori, dei bambini. Durante lo svolgimento delle attività della Commissione sono state sentite altre persone, oltre ai responsabili delle associazioni che si occupano dell'assistenza ai minori. In particolare, sono stati ascoltati, tra gli altri, la direttrice dell'ICAM di Milano, una delle direttrici del DAP, cioè dell'ufficio che si occupa dei detenuti presso il Ministero della giustizia,

assolutamente fronteggiabile con un minimo di buona volontà e con un intervento serio che può essere fatto anche in via immediata: sono 44, infatti, le detenute madri presenti negli istituti italiani, e 45 i bambini

Grazie, ai sette mesi. Di questo stiamo discutendo, Presidente, e dei bambini che subiscono, per effetto di queste permanenze assai brevi, danni gravissimi per la loro salute psicofisica. Di questo parliamo.

tutti ci siamo resi conto - ce l'hanno sottolineato anche gli esperti che abbiamo audito - che ovviamente non è possibile mettere i detenuti padri nelle sezioni a custodia attenuata previste per le detenute madri. Quindi è necessario che vengano allestite allestite apposite sezioni specializzate, altrimenti questa parità di generi, che in questo caso serve ad assicurare dei diritti ad alcuni minori, non si potrà realizzare mai.

in questa situazione è perfettamente praticabile da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Ministro della giustizia dare una risposta al problema.

Capigruppo. Sono trascorse più di due ore da quando abbiamo posto l'esigenza di sapere se il ministro Maroni intende venire in quest'Aula a riferire,

totale contrarietà alla tecnica dei "pianisti", tanto a destra quanto a sinistra di questo emiciclo, desidero segnalare un abuso d'ufficio commesso poco fa in quest'Aula quando è stata ritirata la mia tessera, che non aveva espresso alcun voto. Nessuno può essere autorizzato a ritirare le tessere dei senatori là dove non ci sia stata espressione di voto, e poiché nessuno dei miei colleghi è autorizzato a votare al mio posto, prego il Presidente, nelle prossime occasioni, di non far ritirare la mia tessera se non risulta un voto fantasma. Se sono presente voto, se non sono presente non voto, ma la mia tessera rimane al suo posto e non deve esserci alcun

stata accettata l'idea di attendere la lettura del calendario perché rispettosamente in attesa di una notizia da parte del Ministro, ma credo che il tempo ormai sia tale da costringerci a fare questa discussione. La pregherei pertanto di dirci come intende procedere.

mi permetto di eccepire alcune affermazioni fatte poco fa dal senatore Benedetti Valentini, non relativamente al buonsenso, perché si tratta di opinioni, chiaramente, ma in relazione ad alcuni fatti.

Sono di ritorno dall'ICAM di Milano: tutto ciò di cui abbiamo discusso all'interno della Commissione, ma anche durante il primo dibattito generale, oggi avviene. Allora mi domando: perché

Dal numero di 58 detenute di quest'estate si è arrivati al numero di 46 di due settimane fa. Può darsi che si sia abbassato il tasso di criminalità in Italia. Io ritengo sia così, ma a sentire la maggioranza siamo assaliti dai rom e dagli immigrati, e quindi, molto probabilmente, c'è un'emergenza, ancora una volta,

vorrei ribadire al senatore Benedetti Valentini che noi siamo ben consapevoli dell'esistenza dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, n. 354, che consente al giudice di autorizzare, se ne sussistono le condizioni, un detenuto a recarsi al capezzale di un familiare che sta morendo. Ma qui la situazione è diversa. Noi diciamo che, fermo restando questo potere, che resta intatto nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, si vuole attribuire a un bambino, quindi a un minore che si trovi in ospedale e versi in pericolo di vita, ossia in condizioni gravissime, oppure che si trovi in ospedale per una malattia gravissima, la possibilità di essere assistito dalla madre o, se questa è impossibilitata o è morta, dal padre. Si tratta quindi del riconoscimento di un diritto umano, fondamentale nel rapporto Grazie, che molto probabilmente morirà o è affetto da una malattia gravissima. Questo è il senso dell'emendamento. Si prevede naturalmente che il giudice possa avere delle valutazioni discrezionali quando sia stata sospesa la patria potestà ovvero quando il minore sia stato affidato ad altri, per cui è la posizione del minore su cui si incentra l'interesse di questo emendamento.

la permanenza ospedaliera o comunque la grave malattia del minore, in maniera che ben si comprenda la ragione di questa norma.

Non si comprende per quali motivi, rispetto ad una popolazione di 44 detenute - non credo che tutti i figli di queste detenute siano in pericolo di vita o siano affetti da malattia gravissima non si possa consentire ad un minore di potersi giovare dell'assistenza della madre o, quando questa è morta o è impossibilitata a farlo, del padre. Madre e padre - ripeto rispetto ai quali non sussistono cause di incompatibilità, perché è evidente che nessuno vuole mandare al capezzale del minore magari un padre che abusava del figlio. Ma vogliamo prendere

Presidente, non sarà un Paese civile. Noi vogliamo vivere in un Paese civile, e questo si può fare: ripeto, stiamo parlando di un campione di detenuti esiguo e non di una popolazione estesa rispetto alla quale

questa espressione - per cercare di sanare un danno che il bambino vive non per colpa sua, ma per piena e consapevole responsabilità del genitore. Nel momento in cui il bambino è ammalato, e soprattutto se è in pericolo di vita, si crea un'ulteriore situazione di danno: la relazione madre‑figlio e padre‑figlio ma soprattutto madre-figlio, nel momento in cui il figlio è piccolo, quando vive una situazione di gravità delle sue condizioni di salute, è essenziale, anche per la ripresa delle condizioni stesse. Quindi, trasformare il diritto di visita in diritto di assistenza (quello che prevedono i prossimi emendamenti) credo che sia in in profondissima sintonia, ed è come se fosse parte integrante di questo disegno di legge, è nella sua *ratio*. Ora, siccome non si vuole modificare nulla,

pur non approvandolo, su questo emendamento, assumendosi però la responsabilità in un prossimo - immediato, spero - provvedimento di modificare questa norma. Altrimenti, noi approviamo una legge che è buona, valida, saggia nei principi, ma che contiene una norma che è in contraddizione con la stessa *ratio* legislativa.

Quindi, credo che l'assunzione da parte della maggioranza di questo impegno sia il minimo che oggi possiamo chiedere nel momento in cui approviamo questa legge.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato, a maggioranza, modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 7 aprile. Per questa settimana restano confermati gli argomenti già previsti in calendario. Per quanto riguarda il disegno di legge recante modifiche al codice di procedura penale a tutela del rapporto tra detenute madre e figli minori, i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi al fine di pervenire al voto finale entro la seduta antimeridiana di domani, per la quale non è previsto l'orario di chiusura. Inoltre, la seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 20,30, anziché alle ore 20 come precedentemente stabilito. La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, verranno esaminati il disegno di legge concernente l'abrogazione dell'equipollenza tra laurea in scienze motorie e laurea in fisioterapia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nonché il disegno di legge riguardante il contributo previdenziale integrativo per gli esercenti attività libero-professionali, già approvato dalla Camera dei deputati. Saranno inoltre discusse la mozione Baio sui presidi diabetici, nonché la mozione Bianconi sulla diagnosi e la cura del tumore alla mammella. Nel pomeriggio di giovedì 7 aprile si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre chiesto la disponibilità dei ministri Maroni e Galan per riferire rispettivamente sui flussi migratori a Lampedusa e sulla politica dei beni culturali. Signora Presidente, onorevoli colleghi, nella Conferenza dei Capigruppo il Presidente del Gruppo dell'Italia dei Valori non ha approvato questo calendario

quest'Aula ha esaminato i disegni di legge nn. 804 e 841 relativi all'istituzione delle squadre investigative comuni sovranazionali. Non si poté pervenire al voto in quanto mancava la relazione tecnica del Ministero della giustizia.

Devo denunziare che questa situazione si sta ripetendo su altre materie. Dal mese di ottobre, nelle Commissioni 1a e 2a non vengono forniti pareri del Governo sul provvedimento in materia di corruzione (ossia sei mesi per fornire pareri su emendamenti).

in quanto il Governo non poteva esprimere il parere su un ordine del giorno. Non è pensabile che ci sia da parte del Governo questa lentezza esasperante. Il Governo dica se alcuni provvedimenti li vuole portare avanti oppure no *(Applausi* *dal Gruppo IdV)*: le squadre investigative sovranazionali

a causa delle quali fu fatto un Consiglio dei ministri straordinario provocando il legittimo impedimento del Presidente del Consiglio nel 2010 (processo Mills) perché era necessario intervenire sulla corruzione, dopo sei mesi aspettiamo ancora i pareri del Governo sugli emendamenti. Noi chiediamo che il Governo sia rispettoso del Parlamento e per questo motivo, per quanto oggi ci riguarda, chiediamo che l'Aula difenda le proprie prerogative votando come modifica al calendario dei lavori l'introduzione dell'esame e votazione dei disegni di legge nn. 804 e 841 che abbiamo già discusso. Vi esorto a difendere le nostre prerogative dinanzi ad un Governo che in alcune situazioni è troppo lento e va sollecitato.

e votare. Se il Governo si degnasse di dare qualche risposta, visto che fino ad oggi non lo ha fatto, saremmo lieti di votare il calendario stilato dalla Conferenza dei Capigruppo. Oltre a questa questione, signora Presidente, che molto opportunamente è stata sollevata dai colleghi dell'Italia dei Valori, ve ne sono altre due, parimenti gravi, la prima delle quali riguarda la circostanza che il nostro Gruppo parlamentare da circa tre settimane chiede la calendarizzazione di una mozione sul ripristino delle risorse che riguardano il Ministero dei beni culturali e che hanno determinato le dimissioni del presidente del Consiglio superiore dei beni culturali. Prima ci è stato detto che questa mozione non poteva essere discussa perché il Ministro dai giornali avevamo appreso, noi e la maggioranza - forse si sarebbe dimesso. Poi si è dimesso, ne è stato nominato un altro, e ora ci si dice che non si può discutere perché il nuovo Ministro deve venire a rendere un'informativa al Parlamento su ciò che vuole fare. Questo è un modo cialtronesco di affrontare un problema serio. A questo aggiungo, signora Presidente (se hala bontà di sopportarmi ancora per qualche secondo), che dobbiamo ritenere dalla sua comunicazione che il ministro Maroni non è disponibile, allo stato, a venire questa settimana a riferire in Aula su quello che sta succedendo a Lampedusa, in Sicilia, e sui flussi migratori. L'idea che questo Paese si stia trasformando in una maxitendopoli è una cosa che non desta la preoccupazione del Governo, che non intende venire in Aula a spiegarci cosa intende fare. Apprendiamo da un'agenzia che il Consiglio dei ministri straordinario, epocale, convocato per domani per affrontare questi temi, è stato rinviato a giovedì.

dal Governo, che abbia prodotto uno straccio di effetto su Lampedusa, sulla Sicilia e in qualsiasi altra parte del territorio nazionale. Tranne qualche battuta oscena del ministro Bossi, dal Governo non abbiamo avuto dal Governo alcun segnale di esistenza in vita. Questo è estremamente grave ed oggettivamente

con le comunicazioni del Governo sulla situazione a Lampedusa e sui problemi dell'integrazione.

tecnica e la presenterà? Oppure continuiamo a mettere all'ordine del giorno, senza poterli votare, questi provvedimenti, condivisi da tutto il Parlamento?

il piano di evacuazione; quali sono i siti che sull'intero territorio nazionale accoglieranno gli immigrati, quelli già giunti e quelli che ancora giungeranno; perché è stato attivato in modo assolutamente unilaterale, senza concordarlo né con le popolazioni locali né con il governo regionale, il centro di Mineo, dove si sta consumando una commistione impropria tra richiedenti asilo ed immigrati; perché continua ad essere chiuso l'aeroporto di Trapani-Birgi, così mettendo in ginocchio l'economia di una provincia vocata al turismo. Domando perché

segnalando che il Governo non aveva provveduto a coprire le esigenze finanziarie riguardanti la costituzione delle squadre investigative sovranazionali. Se anche domani mattina mancherà la relazione, che il Senato metta all'ordine del giorno questo punto è del tutto inutile e sarà ancora una volta una presa in giro dell'attività del Senato da parte del Governo.

Signora Presidente, noi voteremo contro la richiesta di modifica del calendario proposta dal senatore D'Alia. A noi spiace constatare come i colleghi senatori siciliani

alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Credo che il Governo non possa rimanere indifferente soprattutto agli insulti e agli epiteti che sono stati rivolti ad autorevoli Ministri e membri dell'Esecutivo, perché la dialettica politica è un conto, e l'insulto personale che abbiamo sentito è un altro conto! Aggiungo che siamo di fronte ad un'emergenza determinata da una guerra in corso dall'altra parte del Mar Se volete che non usi il termine «guerra», potrei definirla un'operazione di pace internazionale che però purtroppo deve ricorrere anche a strumenti di guerra, a bombardamenti e così via. Per tale situazione

alcune sbrigative soluzioni che passano attraverso il mettere a rischio la vita di coloro che cercano di venire in Italia non sono praticabili. Quindi, la prima cosa che fa il Governo è quella di cercare di salvare la vita a coloro che, a torto o a ragione, cercano di venire in Italia. Al riguardo ritengo che tutti dovremmo essere d'accordo. Ma non usare, come altri Paesi europei, metodi sbrigativi per impedire l'arrivo di questi migranti, di questi clandestini, di questi profughi - chiamiamoli come vogliamo - vuol dire che da qualche parte devono sbarcare e allora nasce il problema drammatico di Lampedusa, in prima linea e non può farsi carico di quel carico umano, dolente, che cerca salvezza in Italia. Ma allora, se non possono stare a Lampedusa, da qualche altra parte bisogna portarli. Non mi sembra però, dalle parole di alcuni colleghi,

Quando ho ascoltato il richiamo, giusto, secondo cui il Governo deve farsi carico in queste ore dei rapporti internazionali cercando di parlare con i governanti della Tunisia,

Le stanno chiedendo di rispondere sul calendario. Non entri nel merito delle questioni se è possibile. Colleghi, per cortesia, la Presidenza è stata chiara. Portate pazienza. Signor

Senatore Garraffa, la richiamo formalmente.

collocazioni sul territorio nazionale. L'Italia è ancora un Paese unito. Ci sono 20 Regioni, ma c'è una comunità nazionale...

sta cercando - com'è noto - di collocare fuori da Lampedusa quelli che sono arrivati sull'isola. Ci sono polemiche in corso con alcune Regioni; è giusto che il Governo dialoghi con tutte e 20 le Regioni

e Stato, tutti sullo stesso piano per farsi carico dei problemi senza alcuna subordinazione gerarchica, il Governo, che attualmente sta dialogando con tutte queste componenti, ben volentieri verrà anche in Senato. Verrà il ministro Maroni...

tenendo conto che in queste ore, per questa emergenza, il Governo è impegnato su più fronti, come lo dovrebbero essere anche Comuni, Province e Regioni che fanno parte della stessa Repubblica.

però qui noi abbiamo chiesto solo ed esclusivamente di votare sull'inserimento in calendario dell'informativa del ministro Maroni. Dopo di che, il Sottosegretario, per carità, ha titolo per parlare, ma certamente non per aprire un dibattito su un argomento che non è all'ordine del giorno del Senato non lo è certo non per responsabilità nostra, ma di chi non l'ha voluto inserire sotto la forma dell'informativa che noi stiamo chiedendo. Ebbene, se è così (ed è così, signora Presidente),

Se è così noi ci dichiariamo soddisfatti, però vorremmo capire se è davvero così per manifestare la nostra soddisfazione.

della trattazione dell'argomento di cui abbiamo chiesto di discutere, si presenti qui, entri nel merito, divaghi e non consenta a noi di fare altrettanto, così come abbiamo chiesto. L'atteggiamento del Governo è inaccettabile sotto questo profilo.

del rappresentante del Governo ognuno può avere le sue opinioni, così come sui contenuti. Vorrei però ricordare ai colleghi che la natura stessa del regime parlamentare

che potrebbe anche essere sconveniente nel caso specifico, ma non lo si può regolamentare con i richiami del Presidente o con il Regolamento. In questo modo, infatti, tradiremmo il regime parlamentare stesso e la sua essenza. Quindi, facciamo attenzione a questi aspetti, rientriamo tutti nei ranghi e cerchiamo ora di votare il calendario.

«In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ove non abbia perso la potestà genitoriale,

Sappiamo che una delle altre caratteristiche complicate del nostro pianeta carceri è spesso anche l'assenza di direttori di istituti, in un contesto in cui le nostre carceri sono al di fuori della Costituzione. Noi riteniamo, invece, che un provvedimento del direttore dell'istituto

da parte della madre che si trova in situazione di condanna e, quindi, imputata o internata. Parlo di assurdità del comportamento del Governo perché, quando il disegno di legge è giunto per la prima volta all'esame dell'Aula del Senato,

Tutti avevano acconsentito a un ritorno in Commissione giustizia al fine di poter approfondire alcuni di questi punti. Il Governo stesso si era detto favorevole, in sede di esame degli emendamenti che avevamo presentato avevamo ottenuto diversi pareri favorevoli della relatrice, salvo poi tornare indietro a seguito di pressione e imposizione da parte del Governo.

Sottolineo che si tratta anche di un'assurdità giuridica, perché in questo caso noi chiedevamo di modificare l'articolo e di consentire alla madre condannata di visitare il minore in caso di pericolo di vita;

di civiltà. Va dunque riconosciuto, lo ripeto, il diritto della madre ed il diritto del bimbo. È assurdo che il Governo e la relatrice siano tornati indietro su questo punto, perché se il bimbo è in pericolo di vita, è in pericolo di vita, punto e basta. Colleghi, se votate contro questi emendamenti, votate in maniera disumana.

che serve più la vicinanza e la non solitudine, anche per gli adulti, per guarire meglio e prima,

ospedaliero e si dice che "le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia". Questo significa che di volta in volta la regolamentazione delle visite e quindi di una visita che può perdurare nel tempo viene stabilita dal dal magistrato. Quindi non c'è nessuna negazione dell'ipotesi che la madre stia vicino al bambino, anzi, c'è un'espressa previsione che è un punto di equilibrio fra l'esigenza del bambino di avere la madre accanto a sé in un momento ovviamente difficile e delicato e

che viene lasciata al giudice, e non abbiamo nessuna ragione di non credere che il giudice non darà attuazione a tutti quei principi di umanizzazione che in genere in genere riguardano questo campo delicatissimo. Vorrei portare all'attenzione dei colleghi e delle colleghe dell'Aula alcune osservazioni. In tutti i reparti di pediatria degli ospedali italiani è stata assunta una

aiuta sicuramente per un rapporto di empatia, per un rapporto psicologico, per un rapporto rassicurante; ci sono tanti aspetti che intervengono anche sull'aspetto fisico terapeutico. Se all'interno delle nostre strutture ospedaliere, quelle regolate dalle norme italiane, abbiamo adottato questa norma è perché oggi non solo l'aspetto sanitario, ma anche quello pedagogico ci consiglia di adottare una norma di questo tipo. Quindi, di fronte ad un bambino la cui mamma è detenuta, siamo di fronte ad una situazione particolare. Mi rendo ben conto che non è la normalità dei casi, e magari non avverranno alcuni casi. E allora, perché noi dobbiamo lasciare la decisione all'arbitrio di un giudice? C'è un rapporto di massima fiducia da parte del Parlamento nei confronti della magistratura, però tale decisione non può essere lasciata alla mera discrezionalità. La previsione normativa invece contemplerebbe e raccoglierebbe tutte - dicasi tutte - le osservazioni che la pedagogia contemporanea ci offre e ci mette a disposizione per accompagnare l'accertamento, la diagnosi e la terapia. Soprattutto, e qui ne stiamo parlando, in situazioni di estrema gravità. Porto un esempio per far capire. A qualcuno qui dentro sarà capitato non solo di avere un figlio, perché di figli ne abbiamo tanti e noi non eravamo detenuti o detenute, ma che un figlio abbia avuto un problema urgente, ad esempio un'appendicite acuta che può degenerare in peritonite. Sono questi i casi di gravità in cui è necessario un intervento immediato, senza cadere nella burocrazia giustamente la mamma. Credo che questa norma vada incontro alle nostre giuste, corrette, fondate esigenze di sicurezza,

Non riesco a capire perché: una norma minimale di questo tipo alla Camera dei deputati potrebbe essere approvata, per volontà

Sottosegretario, onorevole relatrice, colleghi, il punto che è stato sollevato è certamente importante. Però la distinzione fondamentale tra assistenza e visita sta nel fatto che

è in fin di vita deve avere accanto il genitore: questo è il punto fondamentale. Poi stabiliamo le norme di sicurezza!

vivendo all'interno del sistema so perfettamente cosa succede quando un detenuto deve ottenere dal magistrato di sorveglianza un di sorveglianza un permesso per uscire dal carcere e recarsi in qualunque posto. Mi rendo conto che nel provvedimento è previsto che il direttore dell'istituto può autorizzare in caso di urgenza il familiare a recarsi a

- delibera in questo senso, significa che il caso è veramente urgente. E se è urgente, non si può togliere al bambino l'assistenza del familiare e limitarla semplicemente ad una visita.

che, ove modificato, ho l'impressione verrebbe messo in un cassetto.

nostro dovere di parlamentari. Non è possibile una cosa di questo genere! Non è possibile pensare che noi dobbiamo a tutti i costi approvare una legge anche se è inutile e, soprattutto, ingiusta.

mai: faremmo una legge inutile, una legge bandiera che non servirà a nulla. Tanto vale lasciare in piedi la legge Finocchiaro, che almeno aveva un suo significato e una sua razionalità. Non dobbiamo per forza intervenire su tutto sbagliando! Non è possibile!

ad essere interpretato da tutti i colleghi della Camera e dalle rassicurazioni che il Sottosegretario preposto ha dato circa la possibilità di visita e, quindi, di assistenza ai bambini sotto ai tre anni.

Noi riteniamo che il tema dell'assistenza ad un bimbo malato sia prevalente e, se la Camera si è distratta, ha fatto altre valutazioni, non è detto che non possiamo concorrere a migliorare il testo, nell'interesse dei minori. Vi invito ancora a riflettere: non è una questione né di destra, né di sinistra; stiamo parlando di bambini che sono in pericolo di vita o che versano in gravi condizioni. *(Applausi dai

Presidente, vorrei rivolgere una domanda ai rappresentanti del Governo. In base alla loro esperienza, che sicuramente non è brevissima, è mai capitato che un provvedimento approvato all'unanimità al Senato, oppure alla Camera, abbia poi conosciuto modifiche migliorative in una successiva lettura alla Camera o al Senato? È quello di cui stiamo parlando. L'incaponimento nel non apportare nessuna modifica, anche quando è evidente l'esigenza di un miglioramento, appare incomprensibile. Altrimenti, diteci che si abolisce il Senato, e risolviamo ogni

il dibattito scambino chi è contrario a questo emendamento per una persona disumana, che vuole impedire alle persone di assistere fanciulli in tenera età in gravi condizioni. O non ve ne importa niente? Ma bisognerà contestare tale opinione, concerne il fatto che il bambino abbia un anno o sei mesi. La norma, così come è nella legge che si appresta a passare, parla di caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore.

l'articolo 30 della legge già vigente prevede che analoghi permessi possono essere concessi, eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità. Questa è già un'ulteriore valvola che assicura la possibilità di contemplare tutti i casi di gravità. È altresì prevista la possibilità, alle condizioni di cui all'articolo 21,

il diritto di visita al minore infermo da parte della madre detenuta. Si tratta, senz'altro, di una positiva e importante novità, ma il testo potrebbe essere ulteriormente migliorato

oltre che di mera visita, della madre al figlio infermo. La nozione stessa di assistenza è più ampia di quella della visita, e consentirà al giudice di modulare di modulare il permesso secondo la durata del ricovero e la gravità delle condizioni del malato. Quindi, il permesso sarà senz'altro non inferiore alla durata del ricovero e non della cessazione della gravità delle condizioni del paziente. Soltanto in questo modo l'articolo 2 avrà effettivamente conseguito dei risultati importanti. Quindi, invito tutti a riflettere e a votare positivamente per tali emendamenti, che hanno questo tenore.

nessun complesso d'inferiorità rispetto all'altra Camera. Crediamo nel bicameralismo, ma non vediamo, in questo caso specifico, la necessità di rischiare di rinviare o, peggio ancora, di bloccare l'approvazione di un provvedimento per di apportare delle modifiche da noi ritenute marginali. Questa non sarà una legge bandiera, non sarà una legge manifesto, ma un importantissimo punto di riferimento affinché l'*iter* di potenziamento e di nuova realizzazione di strutture protette vada avanti nella maniera più celere possibile. Inoltre, noi confidiamo nella giurisprudenza, nella nostra normativa, nella norma di salvaguardia contenuta nel provvedimento stesso ed anche nel buon senso dei giudici e dei direttori nella valutazione dei singoli casi. *(Applausi Quindi non accettiamo lezioni di umanità da nessuno.

in carcere con le loro madri! visto che vi sono 50-60 bambini detenuti ormai da molto tempo. Nel momento in cui l'Assemblea del Senato affronta un tema così rilevante come quello della differenza tra visita ed assistenza o cura,

comprende certamente e il valore di affermare il diritto alla cura nell'interesse superiore del bambino.

Pensate al caso del minore in coma, per il quale la voce del padre o della madre sia ritenuta opportuna per tentare di creare una superficializzazione del coma, ossia un contatto e dunque l'uscita dal coma

no. Stiamo cercando di introdurre il concetto di assistenza proprio per venire incontro ai casi in cui vi è un pericolo di vita per il minore: si tratta di far uscire dal coma un bambino di tre anni che ha bisogno della voce del padre e noi diciamo che questo non è possibile? Ma per favore ragionate,

pensi poi a quanti sono in tutto le donne con i bambini. Ammettiamo che siano 50 e che tutti e 50 i bambini siano in pericolo di vita:

di questa rilevanza e delicatezza. Mancano dieci minuti alla conclusione della seduta, per cui penso sia assolutamente ragionevole disporre in tal senso.

una notizia sugli organi di stampa nazionali che, se fosse vera, ci riempirebbe il cuore di letizia. di uno dei siti di interesse nazionale da assoggettarsi a bonifica, segnatamente l'area di Pioltello-Rodano, un ex polo chimico già oggetto di molte polemiche; il commissario europeo in visita ha il commissario europeo in visita ha dichiarato che la bonifica è stata espletata. A questo punto però non si capisce la notizia di stampa correlata, per cui sarebbe ancora aperta la procedura di infrazione. Delle due l'una: o la bonifica è stata espletata secondo i canoni (e questo doveva avvenire entro il 31 marzo di quest'anno, visto che la Comunità europea aveva concesso una proroga), oppure se contemporaneamente viene detto

come è stato bonificato questo sito di interesse nazionale. Torno a ripetere che la notizia mi riempirebbe di gioia se fosse stato completato l'*iter*, perché si tratterebbe del primo sito di interesse nazionale, identificato dalla legge nazionale, ad essere bonificato.

come riportano sempre notizie di stampa, sarebbe aperto un contenzioso con il precedente titolare della bonifica: titolare che non l'ha espletata e che non aveva neanche versato una fideiussione rispetto agli impegni che aveva assunto. Ora, questo è uno dei punti più gravi e delicati dell'accordo che è stato fatto su quest'area. Il

il seguente. L'area è stata bonificata con denaro pubblico; la proprietà - com'era previsto - deve restare agli enti pubblici, che poi faranno, se del caso, la loro variante. Non è pensabile che una persona inadempiente rispetto agli impegni di bonifica, che non ha neanche versato fideiussioni a garanzia della stessa, oggi chieda chieda di essere pagata per dei lavori che dovrebbe aver fatto e che non si è certi che abbia fatto, e per di più rivendichi la proprietà dell'area. Credo che su questo argomento il Ministro debba dare tutta una serie di chiarimenti e di garanzie. Poi, se davvero è stato completato l'*iter* di bonifica dell'area,

Signora Presidente, nella scorsa settimana si sono tenute in varie città d'Italia, e anche in Sicilia, una serie di assemblee dei cosiddetti Vigili del fuoco discontinui. queste assemblee hanno partecipato anche rappresentanti del Parlamento, sia della maggioranza che dell'opposizione. Ritengo sia opportuno, alla luce delle cose che sono state dette e delle promesse che sono state fatte, anche dai rappresentanti della maggioranza, inserire nel calendario dei lavori anche i disegni di legge che darebbero l'opportunità a questi lavoratori di diventare finalmente lavoratori a tempo indeterminato, a prescindere dalla loro condizione e dalla loro età.

si strumentalizzi il rapporto anche politico con questa categoria facendo promesse che poi non vengono assolutamente mantenute. Chiedo, quindi, che nella prossima Conferenza dei capigruppo si possa calendarizzare anche l'esame di questi disegni di legge che giacciono in Parlamento.